L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Come lei ha detto, senatore Peterlini, non può essere vietato di chiedere la verifica del numero legale. È vero che in questa circostanza,

Presidente, l'emendamento 8.207 interviene sui criteri a cui deve attenersi il regolamento che deve essere emanato.

Mi rivolgo al relatore, se mi ascolta: chiediamo che l'esame di specializzazione previsto per il conseguimento del titolo di specialista (una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente) possa essere svolto a livello distrettuale

ai giovani, come sottolineato dal collega Ceccanti, ma anche agli avvocati che hanno acquisito almeno dieci anni di esercizio della professione e che, per il comma 10 dell'articolo 8, dovranno comunque sostenere questo esame.

esprimo parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei seguenti termini: «*Sostituire il comma 5 con il seguente:* «L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale, con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il Consiglio nazionale forense stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità con cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo». *Di conseguenza al comma 4, dopo la parola*«attribuito» *aggiungere le parole*: «e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5» *e quindi, ulteriormente*, *all'articolo 10, comma 2, dopo le parole:* «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista ai sensi dell'articolo 8», *aggiungere le seguenti:* «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

«Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche e sono dispensati, per i primi tre anni, dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6».

mi pare abbastanza evidente che non si possa procedere all'esame dell'articolo 8, in quanto le materie sono fortemente interconnesse. Evidentemente il parere contrario su un emendamento o l'eventuale ritiro - anche parte dell'opposizione - di alcuni emendamenti, qualora altri avessero una valenza che potesse essere per noi convincente, ci imporrebbe dal punto di vista della saggezza giuridica e procedurale di accantonare l'articolo 8 e di procedere

proposti. Perché approvare qualche pezzetto di articolo per poi tornarci su? Francamente non comprendo la posizione del relatore: dia il proprio consenso all'accantonamento e andiamo avanti. Il relatore ha già espresso la sua opinione.

esami dal CNF alla corte d'appello avrà bisogno di una qualche copertura, a meno che non si intenda che tutto questo avvenga senza costi. Esaminare gli emendamenti in questa fase diventa di quello che stiamo facendo in questi giorni: stiamo intrattenendo l'Aula tra una celebrazione e l'altra. La stiamo intrattenendo con la votazione di emendamenti che non si sa

Il relatore è sempre in tempo a cambiare idea - come sottolineava prima il Presidente - e quindi, dopo la votazione di questo emendamento, potrebbe cambiare idea e decidere di accantonare l'intero articolo:

Poi avevamo proposto altri emendamenti di "riduzione" del danno e anche per cercare di collaborare a migliorare il testo Certo è che se ora neanche si sa più quale articolo si potrebbe sopprimere con il nostro emendamento, comprendo che possa essere anche difficile votarlo. Noi infatti chiedevamo la soppressione dell'articolo 8,

appartengono ad un partito chiamato "Popolo della Libertà" la differenza, almeno sul piano delle attività economiche, fra quello che è stato *l'Ancien régime*, quello precedente alla Rivoluzione francese, e un regime di libertà economica, quale quello inaugurato in Europa la legge Le Chapelier del 1791. Il principio cardine della legge Le Chapelier è quello per cui

produzioni nuove, alle produzioni che si collochino in contrasto con il modo tradizionale di svolgere un mestiere, una professione.

un giovane avvocato, o un gruppo di giovani avvocati, si inventi una nuova specializzazione, un nuovo modo di proporre la propria competenza competenza professionale. Con l'articolo 8 voi intendete vietare questa novità; intendete vietare che l'innovazione nel modo di proporsi possa avere corso nel mercato delle prestazioni forensi. Con ciò sostanzialmente sostanzialmente ritornate all'*Ancien régime.* Non per niente questo è il regime che ha tutelato fino ad ora il vecchio modo, il modo tradizionale, di svolgere la professione. Ma in questo modo voi indebolite la professione dell'avvocato

con riformulazioni di emendamenti da parte del relatore o da parte della maggioranza si cambia il regime delle specializzazioni, significa che stiamo ragionando con emendamenti che si riferiscono al testo originario e che potrebbero risultare superati.

delle due strade possibili: o accediamo alla tesi che ha egregiamente illustrato il senatore Ichino, per cui le specializzazioni non devono essere inserite nel nostro ordinamento poiché rappresentano un limite sia per i talenti professionali dei giovani e per il loro sviluppo sia per il mercato,

Questa è la ragione per cui, come già illustrato dal senatore Galperti, nell'emendamento 8.201 noi prevediamo che la specializzazione professionale sia una «specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale

inoltre che, potendo derivare dall'acquisizione o meno del titolo di specializzazione delle conseguenze sulla vita dell'avvocato e comunque la possibilità di non potersi iscrivere a determinati albi e di non esercitare, per esempio, l'attività di difensore d'ufficio, questa specializzazione - che ricade così seriamente anche sulla vita dell'attività giudiziaria, oltre che sul mercato e su un'attività stragiudiziale in generale - debba essere determinata con regolamento approvato non dal CNF anche per evitare il solito conflitto nelle funzioni e nelle attribuzioni del CNF, che da una parte regolamenta la vita degli iscritti ai consigli degli ordini territoriali e incide sulla loro iscrizione e cancellazione all'albo

delle associazioni maggiormente rappresentative, ma anche acquisendo - voglio spiegare bene perché parlo di acquisizione di pareri - il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario

è vincolante; è tuttavia un parere e non possiamo cambiare la natura degli atti, né la natura e le funzioni degli organi di rilevanza costituzionale. Il senatore Ceccanti è intervenuto spiegando anche la necessità che le specializzazioni siano, tra l'altro, tali da consentire l'esplicazione dei talenti, da non limitare i giovani avvocati e naturalmente da riconoscere e naturalmente da riconoscere anche associazioni specialistiche nel rispetto di determinati requisiti, come ha ben chiarito ieri il senatore Galperti,

non possano accedere alle specializzazioni o abbiano delle limitazioni e che comunque, se si vogliono specializzare, si debbano sottoporre

già da 10 anni. Il comma 10 dell'articolo 8 crea infatti un conflitto tra generazioni e non trova nessuna giustificazione nemmeno a livello costituzionale. Per questo insisto per l'accoglimento dell'emendamento

si creano meccanismi di controllo sugli iscritti agli ordini forensi e si cerca di imporre la supervisione degli anziani sui giovani. Infatti, il potere che viene dato ai consigli dell'ordine e al CNF proprio in merito alla specializzazione degli avvocati, nei fatti,

la formazione e l'aggiornamento che loro stessi - consigli dell'ordine, CNF, in sostanza avvocati già affermati - disciplinano, decidono, istituiscono, prescrivono e sanzionano anche disciplinarmente,

poi per lui gestisce, supervisiona ed amministra corsi, ovviamente a pagamento. Dunque, è un altro modo per conferire compiti a chi controlla le libere professioni

sempre attuale ed in evoluzione, ad indicare la tipologia di legali di cui ha bisogno il cittadino e, di conseguenza, a creare specializzazioni e competenze di volta in volta, non perchè istituzionalizzate o bollate con il timbro degli ordini stessi, del

a ciò che gli anziani mirano ad evitare imponendo la formazione dei *senior*. Infatti, possono specializzarsi solo avvocati iscritti all'ordine da almeno quattro anni. L'autoreferenzialità prevede perfino che sia il regolamento

con il quale si chiede di sopprimere le parole «e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9» e conseguentemente di sopprimere il comma 9,

che non siano sentite le associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo,

il comma 9 di cui lei chiede la soppressione è così formulato: «Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale».

Vede, senatrice, esistono già da decenni le associazioni specialistiche degli avvocati, alcune delle quali - come le camere penali - hanno riconoscimento anche normativo. parlare tanto per parlare di tutto e non parlare dell'emendamento a me sembra un fuor d'opera.

ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni».

in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale» per le specializzazioni dei «percorsi formativi e professionali»

scriverlo nella legge, a nostro avviso, non ha alcun senso. Quindi, con l'emendamento 8.208 si intende sopprimere le parole «di durata almeno biennale».

vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Corte di giustizia europea ha ripetutamente sancito che, nel porre requisiti di anzianità continuativa e ininterrotta, ad esempio ai fini di promozioni automatiche, di itinerari di carriera e di altri benefici simili, si pone in essere una discriminazione indiretta nei confronti delle donne: è infatti noto che nell'attività lavorativa delle donne le interruzioni sono più frequenti rispetto a quella degli uomini, per ragioni

legge a questa giurisprudenza della Corte di giustizia europea, evitando che la norma assuma il connotato di una discriminazione indiretta ai danni delle avvocate, le quali potrebbero avere

del muro impermeabile, ermetico a qualsiasi osservazione che viene dall'opposizione, per considerare l'opportunità di evitare questa violazione del diritto comunitario.

della legislazione ridondante, non debba anche occuparsi di farli in qualche caso preventivamente e se il Governo non debba intervenire sulla qualità della legislazione.

dell'impossibilità di parlare utilmente in quest'Aula degli argomenti che interessano i nostri concittadini. Il mondo si interroga su una crisi finanziaria grave, sulle misure che si devono prendere

alla qualità normativa. Il Governo ha previsto un Ministro per la semplificazione che ogni tanto fa degli *show* per dire che si aboliscono delle leggi che di fatto non funzionano più, non esistono e che sono desuete, mentre dovrebbe occuparsi seriamente di concorrere all'attività legislativa anche con i suoi pareri per evitare per evitare che la normazione che si fa oggi sia destinata ad aggravare in un modo insostenibile la vita del cittadino, delle imprese, dei professionisti e in generale il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. È un tema serio, signora Presidente, nel momento in cui ci accingiamo a votare l'articolo 8 di questo disegno di legge, formato da

non è detto che l'affronti come facciamo noi. Forse questo dibattito, colleghi, che stiamo svolgendo ci interpella sulla qualità e la natura dei dibattiti nell'Aula del Senato, perché penso che - ne parlavo col collega Follini e prendo a prestito un suo argomento, e concludo quando il ministro Tremonti va a fare un'importante comunicazione sulla crisi economica e le decisioni che il Governo italiano ha preso assieme ai Governi europei su misure che preoccupano tutti i nostri concittadini, forse il Senato della Repubblica dovrebbe porsi il problema di invitarlo qui e di garantire che, anziché i 40 deputati che c'erano alla Camera, ci siano 200 senatori, per dimostrare che questo è un luogo nel quale non soltanto si fa una legislazione di dettaglio frustrante, destinata ad essere ulteriormente rivista e magari finire su un binario morto, ma un'attività significativa, coerente con l'impegno che ognuno di noi ha preso con gli elettori, cioè di essere qua a rappresentarli e servire il nostro Paese. Non è quello, signora Presidente, che stiamo facendo con un tipo di normativa di dettaglio, snervante come quella che stiamo affondando. Quindi, la mia dichiarazione di voto, perdonatemi, è piuttosto una testimonianza schietta ai colleghi sull'organizzazione dei nostri lavori e sull'impossibilità di prendere in giro gli italiani sulla semplificazione legislativa, quando il nostro lavoro è di complicazione legislativa. Senatore Rutelli, capisco che questo argomento è provocatorio da parte sua, però, a me pare che sia diverso il concetto di semplificazione che sta alla base di un Ministero che vuole eliminare delle norme inutili e ormai superate. Lei fa riferimento ad un articolato e ad una norma che è stata costruita così in Commissione con l'apporto di tutte le forze politiche, perché noi siamo partiti da un testo che esce da un Comitato ristretto. Allora, nel concetto di semplificazione che lei adesso sta richiamando, non vorrei che finisse per identificare invece una banalizzazione, che non è quello che noi vogliamo fare, perché stiamo affrontando un tema, quale quello delle specializzazioni dell'attività professionale di avvocato, che è nuovo, e come tale va dettagliato. Mi pare che questa fosse stata anche l'idea di tutta la Commissione, nel momento in cui è andata ad elaborare un testo che potrà essere anche discutibile e in alcune parti non condiviso, ma che deve essere apprezzato proprio in quel dettaglio,

rispondere anche all'obiezione che noi abbiamo mosso circa il requisito della continuità e del carattere ininterrotto dell'anzianità di esercizio della professione. Quest'ultimo - ripeto - è un requisito che la Corte di giustizia delle Comunità europee non ammette, e a cui la la Corte stessa riconnette automaticamente un connotato indirettamente discriminatorio nei confronti delle donne. Questo vale non solo per un termine di quattro anni, ma anche per un termine di un anno: la Corte non fa differenza. E, d'altra non si vede il motivo, la ragion d'essere e l'interesse a cui risponde un requisito di questo genere, salvo quello di rendere più difficile l'accesso a una specializzazione o a una qualifica professionale. Non si capisce a *pro* di chi, se non a difesa dei vecchi.

la mia considerazione si può riassumere in un concetto molto semplice. Noi non stiamo facendo una legge: stiamo facendo un regolamento. Se lei va a vedere, noi stiamo dettando le linee di dettaglio che regolamentano un'attività così importante tra le professioni italiane. Io penso invece che, quando parliamo di qualità della legislazione, dobbiamo chiarire che il Parlamento fa una legge in cui detta gli indirizzi, ma non non deve adottare anche i regolamenti. Il livello di dettaglio folle di questa normativa indica, signora Presidente, che stiamo facendo piuttosto un regolamento attuativo che non una normativa di carattere generale.

Perché, se la ragione di questi emendamenti risiede nella proposta che ha avanzato il senatore Ichino, allora la loro formulazione è sbagliata. Sarebbe bastato introdurre la precisazione che il senatore Ichino ha fatto;

delle specializzazioni - quindi di un tasso ulteriormente alto di qualità all'interno della professione forense - e di un regolamento dettato dal Consiglio nazionale forense e stiamo assegnando i paletti che il Consiglio nazionale forense dovrà rispettare nel momento in cui emanerà quel regolamento.

vi sono precedenti in materia: la Cassa nazionale di previdenza attribuisce alle avvocate madri una serie di attenzioni, dovute e riconosciute da molteplici anni, equiparate a quelle di alti livelli di lavoro dipendente)

ci troveremmo paradossalmente ad affrontare un argomento altamente qualitativo come è la specializzazione in un contesto in cui chiunque e indipendentemente dal numero degli anni, stavolta sì interrotti o sospesi, potrebbe parteciparvi. In sostanza, signora Presidente, e io mi avviassi ad avere un ulteriore titolo nei confronti della clientela dicendo: «Ho studiato, sono preparato, sono formato maggiormente in una determinata per accedere a quel corso e poi sostenere il relativo esame ho impiegato 10, 15 o 20 anni. Ecco perché tali emendamenti sono sbagliati, per la loro formulazione e perché inducono evidentemente in errore rispetto alla bontà dell'obiettivo iniziale.

perché il fatto di essere donna, madre, avvocato e anche specialista mi dà una sensibilità particolare al tema che egli ha affrontato.

Vorrei semplicemente ricordare che in questo caso si sta parlando dei corsi di specializzazione, i quali hanno evidentemente un duplice contenuto, di natura semplicemente didattico-dottrinaria e di natura pratica. Non è detto che necessariamente tutte le facoltà di giurisprudenza siano automaticamente in grado di erogare questo genere di corsi, soltanto alla formazione da un punto di vista scolastico, ma anche all'esercizio specialistico di una branca professionale. Ciò significa che necessariamente le singole facoltà dovrebbero in qualche modo attrezzarsi anche per quanto riguarda gli aspetti pratici dello svolgimento dell'attività di specialista. Questa è la ragione per cui necessariamente le abbiamo ricomprese in questa nozione più generica, prevedendo che potranno tenerli nella misura in cui potranno curare anche gli aspetti di carattere pratico attinenti proprio all'esercizio specialistico di una branca del diritto in senso professionale.

della Commissione bilancio si potrebbe accettare se si scrivesse: «senza ulteriori oneri a carico dello Stato », a meno che non ci diano un'informazione diversa. Dal giudizio espresso dal senatore Mugnai

che le facoltà di giurisprudenza offrono una formazione di carattere dottrinale, ma credo che una collaborazione con le associazioni professionali e forensi, come d'altro canto nel

parere negativo perché ritenevo che quando si faceva riferimento ad «altri enti e istituzioni pubbliche» dovessero essere ricomprese anche le facoltà di giurisprudenza. Gli argomenti che ha trattato il senatore Saccomanno e l'indicazione del senatore Valditara di rimodulare l'emendamento

la Commissione bilancio aveva dato parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che fosse inserita la medesima clausola d'invarianza finanziaria già espressa sulla norma del testo.

la lettera *e)*, che recita: «i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni».

ma semplicemente perché sono iscritti all'Albo da almeno dieci anni. Tutto questo, fra l'altro, si inserisce nell'autoreferenzialità, perché non è soltanto il requisito meramente tecnico di essere iscritti all'Albo da almeno dieci anni,

Camere penali che sostengono l'utilità delle specializzazioni: «La specializzazione forense è uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire la qualità della prestazione professionale; non è tollerabile che sia legittimata l'autocertificazione di specialista in più settori del diritto senza alcun controllo di qualità. Quale sarebbe la reazione dei cittadini se il Parlamento consentisse Il diritto di difesa è un bene primario, come il diritto alla salute, e rispetto ad esso lo Stato non può consentire inganni ai danni dei cittadini, al solo fine di di mantenere la rendita di posizione di coloro che, in assenza di una regolamentazione della specializzazione, si sono abituati a vendere un inesistente sapere in ogni branca del diritto».

Presidente, mi duole rilevarlo, ma io ero qui in Aula: non ho avuto il tempo materiale di premere il pulsante.

parte, se la verifica del numero legale ha un senso, è quello di cercare di agevolare i lavori laddove i parlamentari sono in Aula. Questo è anche il senso di quel minimo di tolleranza che è sempre stato consentito. A volte la tolleranza la tolleranza è anche troppa, in questo caso - mi permetta di rilevarlo - c'è stato un atteggiamento eccessivamente categorico. Io le chiederei di ripetere la votazione.

Presidente, rispetto alla storia del Parlamento, è chiaro che questa vicenda non comporta modifiche storiche. Proprio per questa ragione, non avendo lei dichiarato aperta la votazione, alcuni colleghi, quali il senatore Pisanu, parlamentare esperto, il senatore Piccone, il senatore Pontone e altri che sono presenti, come si è visto dalla accensione delle luci, non hanno avuto

io vorrei solo che fosse dato atto alla Presidenza che non c'è stato nessun atto di arroganza e che, anzi, la Presidenza si è attivata, con il presidente, per trovare altre soluzioni. Vorrei che mi fosse dato atto di questo.

CASSON *(PD)*. Alla conclusione della seduta odierna, desidero segnalare due situazioni che riguardano i lavoratori.

segnalando la complessità e la difficoltà della situazione, con particolare riferimento alla necessità di tutelare e garantire i posti di lavoro, oltre che la sicurezza della popolazione e dei lavoratori, in una situazione ambientale di fabbrica messa a rischio dai disinvestimenti e dalle mancate manutenzioni.

perché fa riferimento al Fondo per le vittime dell'amianto, costituito con legge n. 244 del dicembre 2007 (legge finanziaria 2008). Sappiamo che ogni anno sono moltissimi gli ex lavoratori che si ammalano di patologie asbesto-correlate e proprio per questo era stato costituito il Fondo, con una dotazione specifica di 30 milioni di euro.

i morti a causa dell'amianto sono almeno 3.000. Credo che sarebbe doveroso da parte del Governo intervenire e dare una risposta a questi lavoratori, che sono soltanto vittime del disinteresse di questo Governo e di questa maggioranza.